«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.20 (testo 2), 2.22 (testo 2), 3-*bis*.l (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 6.55 (testo 2), 3.4 (testo 2), 6.800 (testo 2) e 1.901 (testo 2), esprime parere non ostativo,

della Costituzione, nonché delle proposte 6.800 (testo 2) e 1.901 (testo 2), sulle quali il parere è contrario. A rettifica del parere precedentemente reso sulle proposte 3-*bis*.0.2, 3.0.4,

abbiamo ricevuto un padre, una madre, un fratello e una moglie di soldati israeliani rapiti sul versante del Libano e sul versante di Gaza.

ho riaffermato non solo la nostra solidarietà, ma anche il fattivo impegno del Senato in tutte le sedi, principalmente nella sede propria che è questa, per strumenti parlamentari di indirizzo anche nei confronti del Governo per le iniziative che verranno assunte. La ringrazio, dunque, per averlo ricordato.

È naturale che io prenda atto in modo assolutamente rigoroso dei loro pareri e, in modo particolare, esprima parere contrario su tutti gli emendamenti sui quali il parere è contrario e motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. le chiedo scusa, signor Presidente, se seguirò l'ordine che mi è stato fornito dalla Commissione bilancio. Per questa ragione esprimo parere contrario sull'emendamento 2.20 (testo 2), ma propongo una sua riformulazione

detta data, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366». Si torna, in sostanza, al testo iniziale dell'emendamento votato in Commissione, che aveva ricevuto il parere favorevole da parte della stessa.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.55 (testo 2). Vorrei rettificare l'emendamento 6.800

Per quanto riguarda l'emendamento 6.73 (testo 2) avrei bisogno di un chiarimento e chiedo scusa al presidente Morando, che credo chiamerò in causa.

Vorrei capire in che senso la Commissione ha modificato il proprio parere sul comma 8-*sexies*, cioè vorrei sapere se il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 è diventato un parere contrario semplice oppure un parere favorevole. il motivo di questa domanda, visto che il tema è stato oggetto di particolare discussione. È una questione per me rilevante anche ai fini dell'espressione del parere.

Introduce, cioè, il principio per cui le spese comunali, cioè l'attività dei Comuni che transita attraverso le istituzioni (che sono una forma di organizzazione del Comune) non sono soggette al Patto di stabilità.

senatore Polledri,

il taglio delle tasse alle Regioni. Ministro, lei i soldi li aveva. Lei ha i trasferimenti alle Regioni. Li riallocherà tra qualche mese. Si tratta di ben 3 miliardi di euro. E cosa dite alle Regioni? «Vi diamo il potere di tassare i cittadini». Bel modo di concepire il federalismo. Ma voi i soldi in questo provvedimento li avete trovati.

in esame è previsto un onere di spesa. Non so come si faccia ad ammettere in un provvedimento un differimento termini con conseguente onere di spesa aggiuntivo non previsto nella normativa precedente.

Quando fate il federalismo, avvisateci, perché in qualche modo ci proteggiamo e cerchiamo di metterci in posizione di difesa. Presidente Marino, lei viene dall'America per fare questi disastri? Bisognava per forza prevedere un intervento di questo tipo?

perché lo stiamo votando oggi e soprattutto perché con questo provvedimento non si abolisce il *ticket*: si trasferisce il problema alle Regioni che dovranno sopperire con tassazioni proprie al mantenimento comunque del gettito che questo provvedimento aveva stabilito a livello governativo in 811 milioni di euro. Di conseguenza, non è vero che si toglie il *ticket*, ma si trasferisce il problema alle Regioni. Se poi la spiegazione dell'abolizione di questo *ticket* era di restituire alle Regioni la competenza esclusiva sulla sanità, cioè non un'invadenza dell'articolo 117 della Costituzione, mi domando perché non si è abolito anche quello sul pronto soccorso.

pare oramai evidente che dall'inizio di questa legislatura ci troviamo sempre più spesso in quest'Aula a dover discutere e votare provvedimenti del Governo che si propongono con il requisito della necessità e dell'urgenza, abusando di uno strumento concesso, sì, dalla nostra Costituzione, ma *in primis* al Parlamento eletto dal popolo italiano. Sempre più spesso siamo qui a dover prendere atto di provvedimenti approssimativi e mal congegnati, frutto di scarsa meditazione e scarsa attenzione. Sempre più spesso ci troviamo a dover assistere a tentativi di questa maggioranza di far passare come interesse del Paese dei meri interessi politici e personalistici. Ma ancora più spesso si teme che vi sia un tentativo di instaurare una malsana prassi, di cui avvalersi per correre ai ripari dopo i pasticci combinati dallo stesso Governo. Non possiamo ignorare, di certo, i rilievi già fatti dai nostri colleghi dell'opposizione sull'articolo 1, comma 5, ad uso e consumo di interessi particolaristici nel settore della ricerca, soprattutto nei concorsi pubblici, strumento necessario per attuare quel famoso cambio generazionale posto a giustificazione dell'intervento operato dal famigerato decreto Bersani. Ci chiediamo come sia possibile legittimare agli occhi dell'opinione pubblica e del settore della ricerca scientifica questo tentativo di porre resistenza al necessario cambiamento dei vertici. Non possiamo, infatti, tacere sulla palese inconsistenza e falsità della giustificazione posta nella relazione. Noi del Gruppo della Democrazia Cristiana-Partito per l'Autonomia ci troviamo ancora oggi qui a dover negare il nostro appoggio per l'approvazione di questo provvedimento, ritenuto lesivo della funzionalità del CNR e della sua autonomia, riconosciuta dalla nostra stessa Costituzione e dalla legge. Non riteniamo sussistere i presupposti dell'urgenza per intervenire in graduatorie vecchie di anni o per rallentare l'emanazione di provvedimenti attuativi di provvedimenti di certo da noi non votati, ma comunque ora legge di questo Stato. Non possiamo dare il nostro consenso a un provvedimento che impedisce il ricambio nell'ambito della ricerca, settore da dover valorizzare e rendere più funzionale e non da sclerotizzare ulteriormente. Non possiamo dare il nostro voto a un provvedimento

pur con qualche spazio di miglioramento, ha visto aprirsi delle maglie pericolose in un provvedimento che arriva dalla Camera

quindi, 60 e oltre milioni di euro che non si sa come saranno gestiti). È un modo, signor Presidente, mi consenta di dire, personalistico. È un modo un po'

quindi al punto di vista della trasparenza economica. In quest'Aula ci sono stati poi elementi fortemente peggiorativi, una serie di provvedimenti *ad personam*. Ricordo

se non paga le tasse viene in qualche modo assalito o addirittura deve pagarle in anticipo per centinaia e centinaia di milioni di euro in più di quanto in realtà riceve mentre c'è un'altra categoria di cittadini che hanno beneficiato

basterebbe semplicemente pesare i provvedimenti per vedere a favore di chi sono. Il Parlamento italiano si schiera sempre, metodicamente, a favore del Sud del Paese. Voglio ricordare che il Nord è una parte di questo Paese che

due elementi estremamente gravi: il primo rappresentato dal provvedimento frutto, ovviamente, del ricatto elettorale del *Südtiroler Volkspartei*, che ha deciso di espropriare parte dei risparmiatori italiani di gran parte dei loro *asset*

riescono a trovare 800 milioni di euro per eliminare il *ticket* sulla salute. La tassa sulla salute, come quella sul gioco d'azzardo, è una tassa sui poveri.

MAFFIOLI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006 cosiddetto milleproroghe è stato oggetto di attento esame in Commissione affari costituzionali con un confronto corretto tra maggioranza e opposizione; di questo va dato atto ai componenti della Commissione, ma anche alla disponibilità del relatore, senatore Vitali, e del sottosegretario D'Andrea. Tuttavia, non si possono evitare alcuni giudizi molto critici sui contenuti del provvedimento e su come, ancora una volta, viene utilizzato lo strumento del decreto-legge per «sistemare» alcune situazioni che si sono create grazie all'inerzia del legislatore. Il provvedimento, tra l'altro, tratta di norme che non contengono alcun tipo di proroga e norme dove i termini sono già scaduti e anche abbondantemente. Ci troviamo di fronte a disposizioni che vanno contro le stesse enunciazioni del Governo, che predica rigore e poi non mantiene fede ai propri propositi, a norme che infrangono il diritto sostanziale. Vi sono norme che favoriscono gli amici degli amici o, peggio, parenti stretti del Presidente del Consiglio Tutte le volte vengono enunciati buoni propositi e tutte le volte succede esattamente il contrario, anzi peggio! Ma quando cambierà, finalmente, il modo di governare questa nostra povera Italia? Questo decreto, infatti, tra l'altro, con la formulazione dell'articolo 1, comma 5, prevede che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, i dirigenti degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei precedenti incarichi. Vi sono diversi interrogativi che io ed altri colleghi della Commissione, e non solo, ci siamo posti. Ovvero: come mai tale proroga ostacola lo svolgimento di ulteriori concorsi per l'assunzione di giovani ricercatori? Dove si ravvisa la necessità di questo blocco concorsuale? Dove si ravvisa l'urgenza di questa norma che non proroga termini stabiliti da disposizioni legislative, ma interferisce esclusivamente in provvedimenti interni di un ente di ricerca con una propria autonomia scientifica protetta dall'articolo 33 della Costituzione? Il Governo, se proprio vuole interferire in un istituto di ricerca come il CNR, lo faccia con uno strumento diverso dal decreto-legge! Che dire, poi, quando si legge l'articolo 3, commi 3 e 3-*bis*? Cosa c'entrano con la proroga dei termini? Cosa si proroga? L'articolo in questione, infatti, estende solo l'efficacia di un atto posto in essere tra soggetti privati e cioè tra il consorzio delle cooperative di costruzione e i privati cittadini. All'articolo 4 si introduce una proroga al decreto-legge n. 229 del 2006. A pochi mesi dalla sua approvazione, il decreto Bersani viene modificato. Questo la dice lunga sulla chiarezza di idee di questo Governo e sulla certezza della norma in questo Paese! Ogni giorno si cambia parere. Speriamo di non ritrovarci tra poco a vederci nuovamente sottoposta qualche modifica di norme recentemente approvate. Tra l'altro, la questione è davvero paradossale se si pensa che questo comma prevede la proroga di un termine già scaduto. Si tratta, infatti, del termine fissato dai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in cui si prevede che il termine fissato è di 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge; termine che risulta, quindi, già scaduto poiché detto decreto è stato convertito in legge nello scorso mese di giugno. Come si può prorogare un termine già scaduto? Altri casi: all'articolo 6, comma 1, si riapre un termine già scaduto lo scorso 31 dicembre, prorogandolo fino al 28 febbraio 2007. Sempre all'articolo 6, comma 8-*bis*, si proroga al 31 luglio 2007 un termine scaduto «solamente» il 28 febbraio 1999. Avete capito bene: 28 febbraio 1999! Questo decreto-legge ha assunto la veste di una minifinanziaria attraverso norme che dilatano la spesa e, soprattutto, vanno a toccare quelle previsioni di risparmio della spesa pubblica che dovevano contribuire a risanare l'economia di questo Paese. Rinviare la chiusura di circa 570 organi collegiali della pubblica amministrazione, prevista dal decreto Bersani con 15 milioni di risparmio per il 2006 e 42 milioni a partire dal 2007, dà un colpo sostanziale alle previsioni di rigore per il risanamento della finanza pubblica. Ancora una volta sono state approvate norme in favore di Province autonome e Regioni a Statuto speciale, mentre l'Italia è ricca nel suo territorio di specificità territoriali e culturali che meritano eguale considerazione e rispetto se si vuole realizzare un vero federalismo; norme vergognose che mi auguro siano bocciate dall'Europa. Ancora una volta si è voluto continuare a dare assistenza sociale a rumeni e bulgari, nonostante l'ingresso in Europa di queste Nazioni, senza stabilire un termine a tali interventi, sottraendo così risorse per l'assistenza ad altri immigrati. Si è modificata la normativa relativa al Patto di stabilità, introducendo norme che favoriscono gli enti meno virtuosi, soprattutto in materia di assunzione di personale. Tutto questo mi pare davvero inaccettabile! È questo un provvedimento che, al di là della collaborazione manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo, che ho già sottolineato all'inizio del mio intervento, non può trovare il voto favorevole dell'UDC.

di valore tecnico, spesso anche per norme che hanno un significato rilevante per gli effetti nei confronti dei cittadini.

In questo quadro considero molto positivo l'emendamento che abbiamo approvato che corregge un'incongruenza della finanziaria che riguardava il Patto di stabilità.

che, non avendo sanzioni, potevano esercitare alcuni diritti come le assunzioni a tempo indeterminato. Questo provvedimento corregge un obbligo dei Comuni oggi di poter assumere solo a tempo determinato e quindi è positivo.

La riflessione che vorrei fare è molto semplice: spesso la necessità di proroghe deve essere utilizzata dal Parlamento per avere il senso della difficoltà e della farraginosità

insufficiente, pur avendola appoggiata, la mediazione che si trovò. In proposito, c'è un fatto politico positivo che apprezziamo: il ripensamento delle altre forze dell'Unione sull'obbligo di prevedere un *ticket* di dieci euro sulle prestazioni diagnostiche. In questa stessa Aula avevamo indicato, la senatrice Emprin in particolare, come una misura non solo iniqua, ma dannosa che avrebbe favorito l'esodo dal sistema pubblico a quello privato, com'è di fatto avvenuto con il clamore del mese di gennaio. Una maggiore capacità d'ascolto dei bisogni popolari, che abbiamo rappresentato, eviterebbe il danno invece che ridurlo. Votiamo mal volentieri la proroga, sia pur temporanea, del regime di partecipazione diretta alla spesa sanitaria. Vediamo il rischio che le misure proposte si rivelino ancora una volta inefficaci oltre che inique e per questo continueremo a sollecitare la loro abrogazione in tutte le sedi. Non sottovalutiamo, anzi apprezziamo l'impegno dell'Unione e della ministra Turco volto a superare questo sistema con la prossima finanziaria. Ci saremmo aspettati più coraggio. La verità è una sola:

talune posizioni dure sono giustificate, purché svolte democraticamente, come pensiamo di aver fatto noi. Abbiamo ottenuto qualcosa da questo provvedimento, è inutile dire. Alcune nostre ragioni sono state ascoltate,

chiarendo e spiegando le posizioni di partito su argomenti significativi. Votiamo contro questo provvedimento per tre elementi essenziali, con tre motivazioni. La prima - è già stata ricordata da qualche collega

Nella passata legislatura, e penso anche nell'altra, si diceva che non bisognava mai inserire in un decreto-legge una norma di delega e nemmeno porla nella legge di conversione.

termini sia pure scaduti il giorno prima o lo stesso giorno. Il non rinnovo dei termini costituiva una norma così forte che alcuni disegni di legge, nei quali c'era stata la forzatura per giusti motivi, erano stati rivisti e rinviati all'Aula dal Quirinale.

di Trento e di Bolzano che in questa sede è stato in qualche modo avallato con una decisione che riteniamo pericolosa anche sotto il profilo della dignità del nostro Paese a livello europeo e internazionale. Per questi motivi, voteremo contro il provvedimento

denunciato ciò sia in sede di discussione delle pregiudiziali che di presentazione e discussione degli emendamenti. Si tratta di un provvedimento non omogeneo, nonostante la Camera abbia tanto disquisito sul rispetto delle regole da parte di di questo ramo del Parlamento. Vi sono proroghe scadute su termini scaduti, e quindi non si tratta di vere e proprie proroghe, ma del ripristino di situazioni anteriori con violazioni di diritti acquisiti. Mi riferisco - ad esempio - in particolare alle vicende in materia di espropriazione per pubblica utilità. Si rileva un insieme di invasioni di campo; cito per tutte quelle in materia di

del relatore e all'approfondimento dei temi in campo. Purtroppo, però, devo anche dare atto che il testo licenziato dal Senato è notevolmente peggiorato rispetto a quello della Camera. È peggiorato almeno per tre ragioni: in primo luogo, perché si modificano le norme della finanziaria appena licenziata, inserendo delle eccezioni o delle deroghe al sistema della verifica del Patto di stabilità. Si tratta di due emendamenti molto importanti, uno votato ieri e uno oggi, che pongono grossi problemi per quanto riguarda la coerenza di una scelta politica che sembrava invece ferma e condivisa da parte della maggioranza di centro-sinistra. Diciamo la verità, certi vincoli valgono in eterno per i piccoli, per i figliastri, e invece sono destinati a cadere per i soggetti forti, in questo caso per il sistema delle autonomie. Queste

una presa di posizione rigida da parte del Governo, un allentamento dei freni, e sappiamo quanto incida la spesa degli enti locali sul debito pubblico complessivo. Un'altra questione molto rilevante è quella introdotta in quest'Aula in materia di concessioni per le centrali idroelettriche nelle Province di Trento e Bolzano. Qui non è questione di autonomia delle suddette Province ma si

di carattere applicativo del Regolamento esistente che noi aspettiamo da tempo e che abbiamo invocato, perché così facendo i provvedimenti legislativi, ma anche i decreti‑legge, potranno contenere tutto e il contrario di tutto, in barba alla Costituzione,

unitamente al relatore Vitali e al sottosegretario D'Andrea che hanno realizzato una positiva sinergia per migliorare il testo

i senatori delle aree colpite dal sisma del 1990 (Catania, Ragusa e Siracusa) che hanno avuto la possibilità di chiudere una vicenda contributiva

Presidente, sento il dovere di esprimere, a nome della Commissione, innanzi tutto

e c'era da valutare con molta attenzione la proponibilità degli emendamenti. Si è fatto un lavoro assai rigoroso, come chiestoci esplicitamente dal Presidente del Senato. Desidero ringraziare la Commissione bilancio per la collaborazione che è stata posta in essere, il relatore che si è sobbarcato di un compito così delicato, ma soprattutto, Presidente, tengo ad affermare che in 1a Commissione, nella quale molto spesso ci sono stati scontri molto aspri, si è lavorato notoriamente in un clima di netta differenziazione politica, con uno spirito assai costruttivo di cui hanno dato atto volentieri diversi colleghi. Desidero ringraziare parimenti i colleghi di maggioranza ma ancora più quelli dell'opposizione che ci hanno consentito, in un tempo ragionevole, di esaminare in modo approfondito le questioni che ci sono state assegnate. *(Applausi dei senatori Vitali e Biondi).*

vengono soltanto per votare, facendo finta di non esserci quando si parla delle questioni di loro competenza, come il ministro della giustizia Mastella e il ministro della sanità Turco ieri. Quando si tratta di parlare, preferiscono andare nell'altra Camera. Ciò è spiacevole, nondimeno

il Ministro dell'interno ha già riferito dettagliatamente ieri alla Camera dei deputati ed ha ricostruito quanto avvenuto nell'operazione che nei giorni scorsi ha sgominato importanti cellule terroristiche attive nel Nord del nostro Paese. Il mio intervento, pertanto, costituisce nel suo insieme un secondo tempo rispetto alle comunicazioni del Governo effettuate ieri. Mi consentiranno, quindi, i colleghi senatori di ritornare sugli elementi di fondo delle indagini, ma soprattutto di soffermarmi sugli ultimi sviluppi, avvertendo fin da subito che siamo di fronte ad un'operazione ancora in corso. Mi pare innanzitutto doveroso informare il Senato che nella serata di ieri la Polizia di Stato, coordinata dalla dottoressa Ilda Boccassini, ha scoperto un consistente deposito di armi nelle campagne padovane, dove, durante le indagini, nel corso di pedinamenti degli indagati, gli stessi erano stati visti nell'atto di occultare materiale. Sono stati sequestrati: un fucile mitragliatore *kalashnikov* con relativo caricatore; un mitra Uzi con caricatore; una pistola mitragliatrice Skorpion; una pistola Sig Sauer; una pistola Colt calibro 38; un cannocchiale per fucile; due divise estive della Guardia di finanza; tre giubbotti antiproiettile; varie fondine; una parrucca; numeroso munizionamento di vario calibro, ancora in corso di repertazione. Quanto sequestrato costituisce la dotazione delle cellule milanese e padovana della formazione terroristica. Una dotazione di tutto rilievo che testimonia, da sola, la pericolosità degli arrestati e il grado di efficienza operativa raggiunto. Non vi può essere alcuna sottovalutazione, perché *kalashnikov*, mitragliatori Uzi e Skorpion, oltre a pistole varie, sono, francamente, un po' troppo per essere soltanto l'armamentario di quattro sciagurati. Siamo quindi di fronte ad un'operazione ampia e complessa, che conferma la straordinaria qualità del lavoro investigativo condotto dalla Polizia, a partire dall'agosto del 2004, dal ritrovamento, in uno scantinato di Milano, di materiale di propaganda unito, però, ad oggetti presumibilmente destinati a finalità illegali (passamontagna, *timer* ed altra strumentazione elettronica, attrezzatura tecnica per produrre fiamma ossidrica), e culminato negli arresti dei giorni scorsi. Un'operazione - mi sia consentito dirlo di fronte a questa Camera - da manuale. Siamo di fronte ad un'azione preventiva di eccezionale pregio investigativo: le armi sequestrate il 12 febbraio e quelle rinvenute ieri a Padova avvalorano infatti la considerazione secondo cui, questa volta, siamo giunti, fortunatamente, in anticipo. Voglio anche ricordare che nei tre anni che abbiamo alle spalle l'indagine si è snodata con un controllo pressoché permanente degli indagati senza che, nonostante si trattasse di persone abituate alla semiclandestinità, nessuno di loro si rendesse conto di quanto gli stava accadendo intorno, e questo, ve lo posso garantire, fino al momento della cattura. Nel corso dei servizi di osservazione gli organi di polizia si sono trovati anche nella condizione di rinunciare ad iniziative che potevano risultare intempestive e pregiudicare il disvelamento della più ampia rete terroristica, facendo ricorso al comma 6 dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, 146, che consente, appunto, di differire l'arresto ed altri atti di polizia giudiziaria per assicurare l'ulteriore sviluppo delle indagini in materia di terrorismo e di eversione. Nondimeno si è agito con grande prudenza e mai si sono messe a rischio persone o cose. È il caso del tentativo di autofinanziamento su un bancomat della banca Antonveneta ad Albignasego, in provincia di Padova, che la DIGOS di Padova è riuscita a sventare, il 29 dicembre scorso, senza intervenire, ma attivando a distanza un sistema di allarme appositamente predisposto. Come voi ormai sapete, sono state arrestate 15 persone, tra cui un militante delle vecchie Brigate rosse: Alfredo Davanzo, cinquantenne, già latitante in Francia, poi passato in Svizzera, dove ha iniziato ad operare nella semiclandestinità, infine rientrato in Italia nei mesi scorsi. Sono anche indagate altre 33 persone ed è stata sequestrata una grande mole di materiale: documenti interni, fogli di propaganda clandestina, moltissimo materiale informatico. Tra gli arrestati, oltre a persone già dentro storie di terrorismo, figurano anche giovani non ancora nati quando nel Paese infuriavano gli «anni di piombo». Un numero significativo degli arrestati risulta iscritto alla CGIL. Alcuni fra gli arrestati sono noti come frequentatori del centro sociale Gramigna di Padova. Per tutti l'imputazione è di associazione sovversiva e banda armata; per una parte degli arrestati concorrono reati diversi, fra cui la detenzione illegale di armi comuni e da guerra. In questo quadro, caratterizzato dall'impiego paziente di tutti gli strumenti investigativi previsti dal nostro ordinamento, mi piace sottolineare il prezioso contributo del SISDE, il Servizio informazioni interne, e l'attiva collaborazione degli organi di polizia di altri Paesi in cui sono emersi collegamenti con l'estero. Sono stati documentati, a questo proposito, viaggi di tre degli arrestati in territorio elvetico ove, fin dal novembre 2006, si era rifugiato Davanzo, e dove sono emersi anche contatti con due esponenti dell'estremismo elvetico, fra cui la nota Andrea Stauffacher, animatrice del Soccorso rosso internazionale, il cui studio è stato perquisito, lo stesso 12 febbraio, dalle autorità elvetiche, in esecuzione di una rogatoria internazionale richiesta dalla procura di Milano. Anche la documentazione sequestrata è, oggi, all'esame degli inquirenti. Operazione esemplare, quindi. Quanto è avvenuto testimonia una straordinaria capacità, maturata e consolidata nel tempo, il nostro Paese può essere giustamente orgoglioso. Attraverso l'altrettanto straordinaria collaborazione tra magistratura, polizia e Servizi segreti è stata acquisita una capacità d'indagine e conoscenza del fenomeno assolutamente eccezionale. Un patrimonio che, con eguale determinazione e professionalità, noi intendiamo continuare a impegnare, senza mai abbassare la guardia. Mi pare importante, ora, per la vostra discussione e per le nostre valutazioni, tracciare l'*identikit* ideologico delle persone arrestate. Si tratta di militanti di un'organizzazione terroristica denominata, come vi è noto, «Partito Comunista Politico-Militare», attestata sulle posizioni della cosiddetta «ala movimentista» delle Brigate rosse (detta anche «seconda posizione»), strutturata, in questo caso, a Milano, Padova e Torino. necessario, per rendere più evidenti le mie argomentazioni, fare riferimento alla più volte citata ordinanza di custodia cautelare del dottor Salvini, dalla quale emergono due questioni fondamentali: la prima relativa alla cosiddetta diversificazione tra le «due posizioni» del terrorismo interno, la seconda riguardo il ruolo del bollettino «Aurora», attentamente monitorato in questi anni dalla Polizia e animato dal suddetto Davanzo. Per la prima questione, «Nel 1984 nelle vecchie Brigate rosse in fase di sconfitta e di ritirata dopo la neutralizzazione degli anni precedenti di intere colonne, si erano manifestate, nel corso del dibattito appunto sulla ritirata strategica, due posizioni: la cosiddetta Prima Posizione di impianto prettamente militarista che ribadiva la validità dell'attacco al cuore dello Stato e la Seconda Posizione» - di cui stiamo parlando adesso «che criticava le derive militariste e soggettiviste e sceglieva la linea di una guerra più propriamente rivoluzionaria» - cosiddetta - «di lunga durata (...). Proprio di questa area, molto presente a Parigi, faceva parte Alfredo Davanzo, a lungo latitante in Francia dopo la condanna a lui inflitta dalla corte d'assise di Torino». È in questo quadro che si collocano le pubblicazioni del bollettino. di cui è sicuramente animatore proprio Davanzo, propone la costruzione del Partito Comunista Politico-Militare, secondo il modello maoista della "guerra popolare prolungata" diversificandosi con ciò dal Partito Comunista Combattente, che continuerebbe a dare la prevalenza all'azione militare sull'azione politica di massa, quanto dall'area dei C.A.R.C. e degli altri gruppi radicali antagonisti accusati di attendismo e di aver abbandonato ogni prospettiva realmente rivoluzionaria, sino addirittura a partecipare alcune volte alle competizioni elettorali. Ciò che Aurora propone (...) è l'affiancamento alla propaganda armata, ossia alle attività militari quali attentati dimostrativi ed altro, di un lavoro politico che, inserendosi in situazioni come le lotte sociali in fabbrica, le contestazioni contro le TAV in Val di Susa e le proteste violente nelle periferie, lavori per portare il maggior numero di persone possibile sul terreno rivoluzionario, preparando l'insurrezione ed evitando sconfitte, dovute appunto al soggettivismo, quali quelle subite dalle Brigate rosse che hanno compiuto le azioni contro il professor Biagi e il professor D'Antona».

quando le Brigate rosse arrivarono alla conclusione drammatica e sanguinaria che l'unica opzione che avrebbe consentito il raggiungimento dei loro obiettivi era esclusivamente la lotta armata; a tutti i costi, la lotta armata. Il terrorismo della «seconda posizione» teorizza invece la coniugazione tra lotta armata e scontro sociale. Da qui la necessità della sua presenza nei luoghi del disagio e dell'aggregazione, dove è possibile incontrare, influenzare, condizionare, piegandoli ai propri obiettivi, i movimenti del sociale. Non a caso, dalle telefonate degli indagati emergono indicazioni di lavoro per fare entrare i propri militanti in scuole o fabbriche, luoghi importanti di presenza collettiva. Non vi sfugge che il tentativo di una meno netta separazione e contrapposizione, che caratterizzò invece le Brigate rosse, la cosiddetta «prima posizione», complica l'analisi, costretta a misurarsi con le ambiguità, e legittima la prudenza e l'attenzione con la quale il ministro Amato, a proposito della iscrizione di alcuni arrestati alla CGIL, ha avvertito che può trattarsi «tanto di adesione di questi iscritti alla CGIL a quel gruppo, quanto di infiltrazione della CGIL da parte di quel gruppo». Ipotesi che «entrambe vanno tenute presenti come possibili spiegazioni». Quanto ai segnalati collegamenti con la criminalità organizzata, gli elementi emersi fanno riferimento ad alcuni tentativi di approvvigionamento di armi ed al fatto che uno dei arrestati, Salvatore Scivoli, è anche pregiudicato per rapina, sequestro di persona ed altri gravi reati che ne evidenziano lo spessore criminale. È emerso, a questo proposito, che lo Scivoli aveva fatto cenno alla possibilità, appena avesse raggiunta la disponibilità del denaro necessario, di recarsi in Croazia per acquistare armi ed esplosivi, e proprio ad un esponente della criminalità organizzata nostrana egli si sarebbe rivolto con l'obiettivo di concludere l'operazione clandestina. Il ritrovamento delle armi scoperte ieri rende forse più attuale ed inquietante quella che ieri appariva solo un'ipotesi non realizzata. Gli accertamenti in corso tendono appunto a verificare se vi è stata o meno questa saldatura con la criminalità organizzata e, in caso affermativo, se circoscritta o destinata a sviluppi che per ora non conosciamo. Un capitolo importantissimo dell'indagine riguarda la documentazione probatoria dei programmi terroristici. E' emerso che gli appartenenti al gruppo avevano individuato un'ampia gamma di obiettivi: alcuni oggetto di sopralluoghi, di «inchieste» embrionali; altri solamente ipotizzati in sede di conversazioni intercettate. La solidarietà del Governo e mia personale non può che andare a tutte le persone entrate nel mirino di questo gruppo terroristico. Solidarietà al presidente Berlusconi ed al professor Ichino, ai giornalisti di «Libero», ad altri dirigenti industriali e a quanti lavorano nelle sedi di Sky e Mediaset. Voglio però sottolineare che nessuna delle persone o delle realtà minacciate dai piani terroristici ha mai corso alcun diretto ed immediato pericolo. L'indagine si è sempre curata di garantire la sicurezza delle persone e delle cose che, dalle stesse indagini, risultavano minacciate. E' doveroso aggiungere che questa tutela non solo non è venuta meno con gli arresti del 12 febbraio, ma è anzi stata rinforzata secondo il giudizio e la valutazione dei nostri esperti. Una decisione naturale perché la nostra attenzione è altissima. Nelle ore successive agli arresti, d'altra parte, abbiamo registrato il fatto che attorno al nucleo degli arrestati, quasi a loro protezione, è emerso un reticolo non occasionale di favoreggiamento o di sostegno. Quattro persone sono state arrestate a Milano perché sorprese ad affiggere manifesti di propaganda ed apologia sovversiva nei pressi di una sede CGIL di Sesto San Giovanni. Tra questi c'era Angela Ferretti, compagna di Massimiliano Gaeta, uno degli arrestati del 12 febbraio. un altro elemento: l'azione di polizia si è potuta realizzare, in questo caso, attraverso la felice integrazione fra i servizi di controllo, anche tecnologico, degli ambienti circostanti al gruppo degli arrestati e l'osservazione e l'allarme diretto di un poliziotto libero dal servizio. A parte altri segni di solidarietà con gli arrestati, gravissimo è il gesto intimidatorio contro il dirigente della DIGOS di Padova, contro la cui abitazione si è tentato di appiccare il fuoco con una tanica di benzina. Non sfugge a nessuno in quest'Aula che solo attori non occasionali avrebbero così rapidamente potuto individuare un obiettivo di tale qualità dimostrando di essere in possesso di informazioni sensibili, come l'indirizzo dell'abitazione privata del dirigente della DIGOS. Prima di concludere, vorrei ritornare su alcune questioni di carattere più generale. In primo luogo, vorrei affermare con chiarezza in questa sede che non c'è alcun collegamento tra questa indagine e la manifestazione di Vicenza di sabato prossimo. Nessuno ha mai inteso collegare terrorismo e pacifismo. Né tanto meno lo ha fatto il ministro Amato, come risulta evidente dalle dichiarazioni da lui rese alla Camera. L'impegno del Governo, il compito del Ministero dell'interno e delle forze di polizia è teso ad assicurare che la manifestazione di sabato prossimo possa svolgersi in maniera assolutamente pacifica. L'auspicio che faccio è che questa consapevolezza, ripudiando ogni forma di violenza, sia anche tra coloro che andranno a Vicenza per manifestare le loro legittime posizioni: così funziona una democrazia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, voi sapete che il nostro Paese in passato ha sconfitto il terrorismo degli «anni di piombo». Ho già detto che continuiamo a non abbassare la guardia, né sottovalutiamo ogni pericolo, sia oggi che domani. Non permetteremo però a nessuno, come non lo abbiamo permesso in passato tutti noi, di condizionare la nostra democrazia e la nostra libertà. Siamo una democrazia forte proprio perché siamo capaci di distinguere tra il terrorismo e l'uso della violenza, da una parte, e il dissenso, anche nelle sue forme più estreme, dall'altra. Questa distinzione è fondamentale in una democrazia. Il nostro dibattito, le nostre discussioni devono continuare ad essere ricche ed alimentate dalla diversità. Possiamo permettercelo perché a tutti noi è chiaro il discrimine e il punto invalicabile del confronto anche più acceso e aspro: il rispetto del principio di legalità e mai e in nessun caso l'uso o la minaccia È questo il patrimonio accumulato dalla nostra Repubblica, il lascito ed il retaggio storico delle esperienze che tutti insieme, al di là delle distinzioni, abbiamo attraversato. Non si illudano quanti ancora coltivano il sogno disperato di utopie tragiche: il Parlamento italiano, tutto il Parlamento italiano, la società italiana in tutte le sue articolazioni, il nostro popolo, il popolo italiano, non si farà dividere. La necessità, il bisogno profondo di far barriera contro la violenza conservando l'unità non è patrimonio di qualcuno, ma patrimonio comune rispetto al quale nessuno può vantare primogeniture. Un patrimonio che si fonda sulla concreta esperienza storica di chi ha sconfitto il terrorismo sapendo che quella sconfitta è il frutto, soprattutto, dell'unità e del ripudio di ogni violenza.

Signor Presidente, colleghi senatori, prendo la parola per confermare, a nome del mio Gruppo, che l'appello del ministro Amato e il conseguente intervento del vice ministro Minniti, per quanto ci riguarda, sono destinati a non rimanere lettera morta. Bene ha fatto il guardasigilli Mastella, e bene farebbe l'intera compagine di Governo, soprattutto quei suoi esponenti che hanno provenienze politiche tradizionalmente più «tiepide» verso le divise, a confermare *coram populo* un sostegno forte ed esplicito alle forze dell'ordine, alle forze dell'ordine, alla magistratura e all'intero impianto che sovrintende alla sicurezza del Paese. Il

dicevo, il sollievo per la minaccia sventata non deve allontanarci da una lucida percezione di quanto è accaduto Assistiamo, infatti, ad un risveglio eversivo che il Ministro dell'interno ci ha confermato non essere né isolato, né tanto meno disorganizzato. La replica, dunque, deve essere efficace e senza sconti, e perché sia tale è necessario sgombrare il campo da preconcetti ideologici sul tema, da qualsiasi direzione essi provengano. Va ribadito, una volta per tutte, che il terrorismo non ha colore: sparata da sinistra, oppure da destra, una pallottola produce gli stessi effetti. Il confronto è precisamente in questi termini: la logica della pallottola contro quella della scheda elettorale, del confronto democratico, del pluralismo sociale. Per questo, mentre da un lato ribadisco che l'invito alla maggiore alla maggiore vigilanza interna non deve diventare criminalizzazione del sindacato interessato, dall'altro insisto sulla necessità di far percepire ai tutori dell'ordine che le istituzioni sostengono la loro opera senza «se» e senza «ma». Certamente, i recenti tragici fatti dello stadio di Catania e la riorganizzazione delle Brigate rosse sono contesti molto diversi tra loro. Eppure, tra la morte dell'ispettore Raciti, le scritte infamanti contro la Polizia, il minuto di silenzio profanato dalle reazioni di una tifoseria indegna e infine queste nuove velleità di lotta armata corre in qualche modo un filo rosso di rancore, di diffidenza verso chi serve lo Stato. Si tratta di un legame ammesso con preoccupazione dallo stesso ministro Amato, quando ha stigmatizzato «l'emergere di spunti di ostilità nei confronti delle Forze di polizia». Mai come in questo momento, dunque, le forze dell'ordine devono operare percependo, anche psicologicamente, psicologicamente, il sostegno della società civile e quello di tutti - dico tutti - coloro che la rappresentano nelle Istituzioni. «Stato con la polizia» non vuoi dire «Stato di polizia»: è necessario che qualcuno se lo metta definitivamente in testa o è condannato a vivere da reduce ideologico, proprio come queste Brigate rosse «fuori tempo massimo». Concludo con una considerazione sull'ormai prossima manifestazione di Vicenza. Di fronte alle pur gravi valutazioni del Quirinale, alcuni politici hanno ribadito che la realizzazione dell'evento, come pure la loro personale partecipazione, è scelta imprescindibile di democrazia. Rispetto la posizione dei nostri alleati politici e non mi azzardo ad entrare nel merito delle scelte, ma una piccola considerazione costruttiva vorrei pur farla. Winston Churchill diceva: «Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità, un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà». a livello di compattezza politica del Governo, ma anche e soprattutto di sicurezza pubblica, la contestazione di sabato è più «opportunità» o più «difficoltà»? Il dibattito è aperto. Seguendo la metafora dello statista inglese, io sarei su una linea di moderato pessimismo, ma di certo, in quest'Aula e non solo, c'è chi è ottimista senza alcuna moderazione.

quando ci troviamo di fronte atti terroristici organizzati che mietono vittime tra cittadini inermi, in Paesi in guerra, e che mostrano enormi difficoltà a conquistarsi un confronto parlamentare democratico, la condanna appare comunque scontata. Ma quando questi stessi gesti violenti vengono perpetrati in un Paese come il nostro, che può fregiarsi di una Carta costituzionale tra le più democratiche al mondo e di una legge elettorale come quella in vigore durante la prima Repubblica (che per più di cinquant'anni ha consentito a cittadini di ogni fascia sociale, ma anche a coloro i quali portavano l'ideologia della sovversione, di partecipare alla gestione della *res* *publica*), la condanna è non solo scontata, signor Ministro, ma grave, convinta, senza appello, intellettualmente piena e democraticamente naturale. Uno Stato che sottovaluta, che non presta la dovuta attenzione a questi fenomeni striscianti, che apre la stagione del perdonismo, senza valutare le perplessità delle famiglie dei caduti, è uno Stato che rischia pericolosamente di perdersi nel caos. Non accadde nella prima Repubblica, con la Democrazia Cristiana, il pentapartito e le altre forze politiche che componevano allora l'opposizione (lei lo ha sottolineato); non può accadere oggi, nella seconda Repubblica, di sottovalutare non semplici segnali, ma concretezze, come quelle che abbiamo conosciuto in questi giorni e che lei ci ha sottolineato con il suo discorso. Certo, un sicuro plauso va alla magistratura, ai servizi e alle forze dell'ordine tutte, costantemente in prima linea a contrastare questo fenomeno. Ma oggi, come allora, è la politica che deve affrontare e risolvere il problema in ogni suo aspetto e sfumatura, ma deve farlo ora, subito, prima che decine di giovani, al seguito di cattivi maestri, compiano atti efferati e riprovevoli. Bisogna che il Parlamento si carichi della responsabilità di usare l'arma della prevenzione; una prevenzione basata più sul lavoro, su maggiori certezze per le fasce disagiate, evitando di spargere veleni secondo le teorie della cultura dell'odio, non chiamando mai l'avversario politico nemico, ma uomo o donna che semplicemente hanno opinioni differenti. La prevenzione passa anche dalla consapevolezza che culture diverse possano avere un civile confronto dal quale può scaturire maggior conoscenza e comprensione reciproca. Biagi non ha privato i giovani del proprio futuro e per tale motivo non meritava di certo di essere barbaramente assassinato, ma nessun uomo lo merita. Il suo parere, quello di Biagi, e gli accadimenti successivi lo hanno suffragato. La sua intenzione era quella di aprire con immediatezza il mercato del lavoro alle fasce più giovani. Io e il mio partito, da tempo, portiamo avanti l'opinione che siano sì necessarie maggiori garanzie per i giovani che per la prima volta si affacciano nel mondo del lavoro, ma sempre nell'ambito dell'intuizione del professor Biagi. Per raggiungere un miglioramento di quel provvedimento legislativo non è necessario arrivare ad uccidere. Non si tratta di un atto politico, ma solo di un gesto di ignoranza e di vigliaccheria. La battaglia non deve essere tra le strade a colpi di fucile, ma qui, in questa sede e deve essere una battaglia democratica nell'unico luogo ove le cose possano essere realmente cambiate. Compete allo Stato e al Parlamento ora porre in essere rimedi, privando di argomenti l'estremismo che pesca nel disagio. Tali rimedi passano attraverso intuizioni legislative che consentano alle fasce più deboli di affrontare con maggiore serenità la loro esistenza quotidiana. É, inoltre, demandata agli schieramenti politici la necessità, anzi la responsabilità, di fronte a tali episodi che dilagano nel mondo dello sport e in quello della politica, di abbassare i toni, di sgrossare i propri Masaniello per tentare di rieditare lo stile dei De Gasperi, dei Moro, dei Fanfani, dei Berlinguer, dei Nenni e così via. La politica si riappropri finalmente di se stessa e direttamente dalle mani dei cittadini e non più dalle ricche *lobby* di pressione. Il Parlamento costituisce lo strumento principe della democrazia e allora non facciamo più leggi elettorali che impediscono il suo ingresso nelle sue Aule dove il confronto è padrone. Al Ministro e a questo Governo, con l'appoggio del Parlamento, il compito, quindi, di sradicare alle radici questo vergognoso fenomeno, facendo propria quella responsabilità che fu già propria storicamente dei protagonisti della prima Repubblica. Mai quindi dobbiamo abbassare la guardia di fronte a tali manifestazioni di violenza, ma, al contrario, esse ci devono indurre ad approfondire l'analisi dei fenomeni che vi sono alla base, andando non solo quindi alla ricerca dei colpevoli materiali, ma soprattutto delle cause per poterle rimuovere definitivamente. Tutto ciò è assolutamente necessario in una società come la nostra, che si professa e vuole essere libera, democratica ed attenta all'interesse di ogni suo componente e che vuole prestare la giusta attenzione nei confronti di chi è più debole e privo dei mezzi per poter far sentire la propria voce.

siamo solidi in alcuni convincimenti. Credo sia lo stesso clima registrato ieri alla Camera. Ciò significa che probabilmente, avendone consapevolezza da subito, possiamo fare un buon lavoro in questa direzione. Mi associo ovviamente ai ringraziamenti per la capacità da manuale - com'è stata definita - dimostrata dai nostri servizi, dalla nostra magistratura, dalle nostre Forze di polizia. Entrando nel merito delle comunicazioni che lei ci ha fatto, onorevole Minniti (armi (armi ritrovate stanotte, collegamenti internazionali documentati e confermati, quasi certamente collegamenti con la criminalità comune), credo vi siano tutte le condizioni per dire che ci si trova di fronte ad una cosa seria. Credo vi siano tutte le condizioni per dire che il fenomeno è delle dimensioni in cui é stato rappresentato dai *mass* *media* e non sia da sottovalutare. Credo si debba concordare sul fatto che probabilmente sbaglia in questo caso chi afferma che si tratta di quattro sciagurati. Probabilmente è altro. Probabilmente non ne avevamo consapevolezza. Stiamo lentamente e intelligentemente prendendone coscienza.

il punto di analisi, che si può condividere, è quello del passaggio dalla lotta armata allo scontro sociale, se il punto di discrimine rispetto alle precedenti esperienze è questo, è del tutto evidente che rispetto a questo dato di analisi noi si abbia l'obbligo di essere poi conseguenti nelle decisioni. Lei, signor Vice ministro, ha fatto riferimento alla manifestazione di sabato dicendo che non sfugge a nessuno, e meno che mai all'Italia dei Valori, che non vi è alcuna correlazione. Tuttavia, proprio in relazione a quella manifestazione, noi dell'Italia dei Valori ci eravamo permessi, e lo abbiamo fatto anche oggi, di chiedere soprattutto alle forze di Governo e di maggioranza sobrietà e responsabilità. se siamo di fronte al passaggio dalla lotta armata allo scontro sociale, è del tutto evidente che anche i nostri comportamenti, forse più di quelli di chi oggi è opposizione o minoranza, sono interpretati e leggibili.

Perché non pensare tutti noi che si può manifestare anche non partecipando? Le ACLI hanno trasmesso un loro messaggio alla Nazione, sono presenti sui *mass media*, hanno detto che non vogliono correre il rischio di un ideologismo antiamericano che sembra serpeggiare. Non è anche questo un modo per esprimere le proprie idee, mantenendo manifestando un comportamento che forse da a tutti quanti una mano? Credo sia un esempio sul quale abbiamo il dovere di riflettere anche per il futuro rispetto ad una situazione che non penso ci sfuggirà di mano e che ha però tutte le caratteristiche per essere considerata pesante, importante, vasta, da non sottovalutare. Credo che ogni comportamento

parlamentare che in queste situazioni le forze democratiche debbono e possono avere, e credo avranno. Allora, se così è, per quanto riguarda l'Italia dei Valori, ci troviamo pienamente, ministro Minniti, nei princìpi che ha citato, che sono i princìpi sui quali si sviluppa la nostra democrazia, sia quella parlamentare che quella sociale: il principio della legalità che prevale, prevale, perché è la cornice entro la quale tutti gli altri si vanno ad innescare, e il principio della non violenza. Concludo dicendo che, rispetto a questi principi - mi piace citarlo ancora una volta - quello che ci offrono le ACLI può essere per il futuro un esempio di cui riusciamo a tenere conto in positivo.

signor Vice ministro, il Gruppo Per le Autonomie interviene nel dibattito prima di tutto per esprimere pieno apprezzamento alle parole del Vice ministro e anche a quelle pronunciate dal ministro Amato nella sede della Camera dei deputati. Interviene poi per esprimere il più sentito ringraziamento al lavoro investigativo importante, determinante delle forze di polizia e della magistratura che ci consente oggi di svolgere questo dibattito in un clima preventivo e permette a tutti noi di essere in campo prima che succeda qualcosa di tragico. Questo non è poco e di ciò dobbiamo ringraziare chi da anni - come ci illustrato il Vice ministro - lavora nel silenzio per portare a casa risultati così importanti per le nostre istituzioni, per l'integrità della convivenza civile nel nostro Paese. La nostra solidarietà va anche al dirigente della DIGOS a Padova che, nelle vicinanze della sua abitazione e dei suoi familiari, ha ricevuto un grave atto intimidatorio che, come ha rilevato il Ministro, non è da sottovalutare. Siamo preoccupati per il risorgere di questo fenomeno di cui ancora non cogliamo l'ambito e le dimensioni, che ci riporta a tempi bui che avremmo voluto non rivedere, e di cui, purtroppo, anche in tempi recenti abbiamo visto recrudescenze.

La risposta ancora più che nel passato deve essere trovata tenendo gli occhi ben aperti ai livelli di base delle organizzazioni politiche e sindacali, perché è lì il punto debole, in questo momento di grandi trasformazioni, dove la propaganda eversiva può avere presa facile. massima solidarietà a tutti i destinatari per gli attentati che le Brigate rosse - questi nuovi terroristi - stavano progettando: all'uomo politico, al giuslavorista, ai giornalisti - ripeto ancora - alle forze dell'ordine. La viltà del terrorismo e dell'eversione individua il singolo inerme come emblema del nemico, dell'avversario da abbattere. Ci ricordiamo che il terrorismo ha colpito riformisti come D'Antona, Tarantelli, Ruffilli, Biagi; abbiamo presenti le minacce di questi giorni a Ichino, oltre che al presidente Berlusconi. Coloro, mi riferisco appunto soprattutto alle figure di Ichino e dei riformisti, che si cimentano in questo momento con le grandi trasformazioni della nostra società e con il disagio che queste trasformazioni creano, diventano l'obiettivo di una strategia terroristica che mira appunto ad eliminare quelle persone che queste tensioni e questo disagio tentano di superare con proposte Quindi, il terrorismo non può neppure lontanamente essere giustificato come effetto di quel disagio sociale perché attenta proprio nei confronti di coloro che a quel disagio cercano di dare risposta per superarlo.

nel confronto politico delle possibile ripercussioni negative che l'alzare il livello dello scontro e la demonizzazione dell'avversario possono avere nei confronti di chi vive situazioni di disagio ed è soprattutto in una fascia d'età, come quella dei giovani, dei giovani, che vivono situazioni ancor più difficili dal punto di vista personale. Ci sono, dobbiamo dircelo, forze politiche o meglio parti di forze politiche - mi riferisco a entrambi gli schieramenti - che agitano temi populistici e

Quindi, il no alla violenza, all'annientamento e alla criminalizzazione dell'avversario, ad ogni forma di intolleranza nella vita politica e sindacale, passano prima di tutto attraverso i nostri comportamenti e il nostro linguaggio. Dobbiamo essere capaci di testimoniare nei fatti che la legittimazione di ogni forma di protesta politica passa per il pieno e totale rispetto non solo delle regole democratiche, ma anche dell'avversario.

non è educativo in termini di invito a luoghi di partecipazione e di dibattito politico in cui si dovrebbe insegnare prima di tutto il rispetto dell'avversario e delle regole democratiche del confronto politico.

Governo, onorevoli colleghi, le parole del vice ministro Minniti ci riportano ad un periodo buio per la storia d'Italia che segnò la notte della nostra Repubblica. Anni lontani, ma quanto mai attuali. Quegli anni, definiti «anni di piombo» sono quelli che convenzionalmente vanno dal 1969 al 1989. anni nei quali gli attentati con echi nazionali furono più di 7.000, alcune migliaia i feriti e 455 i caduti, ai quali si aggiungono i più recenti: Massimo D'Antona, Marco Biagi ed Emanuele Petri. Operava in Italia un terrorismo eversivo fatto di attentati, ferimenti, omicidi e stragi. Nel 1979, anno di massima espansione del terrorismo, erano attivi 270 gruppi armati dei quali 215 riconducibili a sigle di sinistra e 55 a sigle di destra. I fatti di questi giorni non ripropongono certo un simile quadro, sia per la forza militare e strutturale della rete eversiva scoperta, sia per il potenziale bacino di connivenza ideologica di cui poteva disporre. È ben diverso - intendo dire - da quell'ampio e diffuso ambito di connivenza e compiacenza che caratterizzò l'eversione ed il terrorismo dei cosiddetti anni di piombo. ciò che ha riferito il vice ministro Minniti è comunque molto grave. L'aspetto inquietante oggi è il filo conduttore che lega alcuni giovani, neobrigatisti, ai vecchi del terrorismo storico. Questo aspetto testimonia, se mai ve ne fosse bisogno, che la storia di quegli anni non è mai stata chiusa, sia per i tanti protagonisti dei quali sono scomparse le tracce, sia per i tanti episodi dei quali non si è mai avuta verità. Un terrorismo quindi che ciclicamente rinasce, un morbo nefasto, che ogni volta che sembra sconfitto si ripropone. Un terrorismo che sembra una sorta di sistema endemico nella nostra società: un cancro, che tuttavia non si può sviluppare in piena autonomia, ma sa trovare spazio nelle contraddizioni gravi e irrisolte del nostro sviluppo economico e sociale, nei fattori irrisolti della nostra democrazia. La straordinaria dimostrazione di competenza ed efficacia che hanno saputo esprimere in questi giorni la nostra polizia e la nostra magistratura certamente ci inorgoglisce. Ad essi va il nostro sincero apprezzamento e ringraziamento. Ma vi è un aspetto di cui bisogna essere consapevoli: per sconfiggere definitivamente il terrorismo non basta investigare, non basta reprimere; per combattere e vincere il terrorismo occorre saper trasmettere in modo profondo democrazia e giustizia sociale. Occorre saper comunicare con i giovani. È necessaria un'azione che, poggiando su verità storiche, sappia fornire alle nuove generazioni strumenti e comportamenti degni di una società civile. Occorre costruire una memoria storica condivisa, che non sia usata, come sovente accade, come una clava nel dibattito politico. Della nostra storia e del filo morale che la contraddistingue dobbiamo avere consapevolezza e memoria, perché i valori che vogliamo affermare devono poter poggiare su basi solide. La memoria e la conoscenza di ciò che c'è dietro a noi e attorno a noi sono quanto di più indispensabile per mobilitare le coscienze attorno ai grandi temi del nostro tempo. Occorre guardare dentro il nostro passato per porre le condizioni affinché il nostro Paese non si ritrovi domani di fronte ad altre possibili tragedie.

Presidente, il nostro Gruppo esprime vera soddisfazione per l'operato della magistratura e delle forze dell'ordine: è stata condotta un'azione preventiva che ha garantito sicurezza nel Paese e ha impedito lo svolgersi di probabili attentati. È la dimostrazione che le istituzioni funzionano e non hanno abbassato la guardia. Il nostro Gruppo esprime anche sincera solidarietà alle società, ai giornali, alle persone e agli uominipolitici minacciati in questi giorni. Signor Presidente, lo facciamo con parole chiare e dirette, senza secondi fini; lo facciamo, ovviamente, non nascondendo le nostre idee. Esprimiamo solidarietà nei confronti del professor Ichino, del quale conosciamo le idee e gli scritti. Egli è considerato, proprio per le sue idee ed i suoi scritti in tema di modifica del mercato del lavoro e dei diritti dei lavoratori, un nemico di questi ultimi. Personalmente ritengo che sia soprattutto una persona che non capisce più le reali condizioni di vita dei lavoratori, le condizioni di lavoro

a tutelare i diritti di tutti, e quindi i diritti del professor Ichino di esprimere le proprie idee e condurre le proprie battaglie, e quelli di chi non condivide, contesta e combatte quelle idee. Credo che questo sia il sale vero della democrazia. Esprimiamo solidarietà al giornale «Libero» e al dottor Feltri, anche se - non abbiamo problemi ad affermarlo - riteniamo che quel giornale esprima una cultura populista, antipolitica, regressiva, chiusa e antieuropea. Ritengo che nelle società moderne e nelle società democratiche debba essere tutelato il bene più prezioso in tema di informazione, cioè la libertà di stampa, anche di chi scrive e professa cose molto distanti da quelle che, personalmente, il mio Gruppo concepisce, così distanti da noi. Anzi, devo dire di più: mi stupisco che l'Ordine dei giornalisti non sia intervenuto su questa vicenda, esprimendo solidarietà a quel giornale.

Berlusconi ha perso le elezioni, se ne deve fare una ragione. Lasci stare collegamenti azzardati e sbagliati tra una sana polemica politica, anche aspra, e il ricorso alla violenza. Non c'entra nulla. La sinistra ha fatto da tempo i conti con il terrorismo. Da questa parte si ricordano troppe vittime della violenza terroristica. Il nostro Gruppo ha una posizione molto chiara al riguardo ed è di chiusura netta. Anzi, qualcuno di noi è pacifista, è non violento, prima ancora che per scelta politica per scelta culturale. È nel nostro DNA. Noi riteniamo che il terrorismo sia la negazione della democrazia, della partecipazione, del confronto, della convivenza. Riteniamo che le indagini debbano fare il loro corso. Auspichiamo che le garanzie giuridiche vengano garantite per tutti, per chi si dichiara innocente, per chi si è già dichiarato prigioniero politico e anche per quelli che hanno pagato il loro debito con la giustizia e ora sono tornati nella società civile. Presidente, ritengo che sconcertino due dati. Il primo è che sono coinvolti i giovanissimi e l'altro è l'iscrizione al sindacato. Ritengo che la questione del coinvolgimento dei giovani forse derivi anche dal fatto che è stato colpita l'ala movimentista delle Brigate rosse, che molto spesso è in contrapposizione con la cosiddetta ala militarista. vi è un problema che ci riguarda tutti, che riguarda l'azione politica e l'azione legislativa, perché questo Paese ha bisogno di fiducia, di futuro, di possibilità di cambiamento; ha bisogno di meno precarietà. è, poi, la questione del sindacato, spesso utilizzato - come, ritengo, in questo caso - come forma di copertura. Capisco la posizione della FIOM che dice di non poter fare l'analisi del sangue a 380.000 iscritti. Tuttavia il sindacato si deve porre il problema di inserire nella propria organizzazione

aspirazioni, sulla volontà di cambiamento della gente. Non vi sono collegamenti tra le grandi iniziative di massa e le azioni di qualche sconsiderato che compie gesti di questo tipo. Credo che chi compia gesti di questo tipo sia fuori dalla società reale, dai problemi veri. Concludo, signor richiamando l'iniziativa di sabato a Vicenza: vi sarà una manifestazione grande, pacifica, una manifestazione di popolo.

significa insultare le persone che con passione difendono il proprio territorio e le proprie idee. Se i terroristi pensano di potervisi infiltrare, troveranno una risposta giusta, negativa, ferma e rigorosa. Signor Vice ministro, attendevamo qualcosa da lei, una relazione che spiegasse un po' all'Aula,

siamo orgogliosi; ma conosciamo le capacità, la dedizione ed anche l'efficacia del nostro sistema delle forze dell'ordine. Abbiamo capito che il fenomeno, forse, è ancora più vasto di quello che l'operazione ha rimarcato; non sono, forse, interessate solo quindici persone,

esempi si danno ai simpatizzanti, ai lettori, ai cittadini e ai giovani, che ascoltano, che guardano, che leggono?

di Feltri, che - guarda caso - ancora in questa sede è stato definito populista, regressivo e avanti con la demonizzazione!). E vengo anche a dire il perché di quest'operazione: appartenenti ad un sindacato non hanno sentito il dovere, in capo al loro segretario generale Epifani, di spendere mezza parola a favore di un giornale che esprime una libera posizione, seppur distante, probabilmente, dal loro sindacato; è stato un gesto di scortesia, sicuramente. Godendo dell'immunità parlamentare che contraddistingue tutti coloro che sono seduti in quest'Aula, posso dire che vi è una complicità morale nel non biasimare questi comportamenti in capo a chi avrebbe dovuto sentirsi corresponsabile, però non vi è stato questo atteggiamento. Quanti esempi abbiamo visto di asprezza oltre il lecito, oltre misura, nel confronto politico, com'è già stato ribadito in qualche intervento in quest'Aula? Ormai non esiste più la contrapposizione, non esiste l'avversario: esiste il nemico. Questi sono i linguaggi che una grossa parte di sinistra ha adottato da tanto tempo. Non voglio esagerare

Bertinotti, che torna dal Chiapas e dice che giustifica le morti e la violenza, perché lì si muore di fame, quindi è giustificato uccidere. Il ministro Ferrero, che nomina come consulente del Ministero un ex brigatista, che pure

Questo è il messaggio che esce. Caruso lo avete fatto eleggere voi in Parlamento. Ha fatto della lotta alle istituzioni la sua ragione di vita, e non mi sembra sia una lotta pacifica quella condotta

Dieci di questi ragazzi, oltre a tutti i dirigenti del nostro partito, sono stati messi sotto inchiesta da un giudice di Verona per delle ipotesi di

Abbiamo riportato abbastanza esempi; a tale proposito, in Aula ogni tanto si cita, non dico a sproposito - bisognerebbe anzi usarlo più spesso - Voltaire. Mi viene da chiedere se ricordano qualcosa degli scritti di quella benemerita persona o se, dopo averli letti, forse sono stati posti in qualche cestino!

non può che portare a ciò, a queste vicende che ci fanno interrogare e ci lasciano con mille punti di domanda. Cosa facciamo oggi? Mettiamo qualche toppa. Il problema è che continuiamo a chiederci cosa si dovrebbe fare

Però, lancio un monito e dico che tutto questo non deve esimere tutta quanta quella parte di sinistra che ho citato in questo intervento a fare un forte e serio esame di coscienza. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto, a nome dell'UDC, esprimo convinto apprezzamento alla relazione che il vice ministro Minniti ha introdotto oggi in Aula al Senato.

Amato. Ma è una relazione alla quale è sottesa una capacità di valutazione e di disegno politico che non può sfuggire all'attenzione di coloro che si accingono, di fronte al riproporsi della fenomenologia terroristica, con molta serietà e con molta gravità. gravità. Accanto all'apprezzamento per la relazione del vice ministro Minniti, un ringraziamento ed un apprezzamento alle Forze di polizia, ai Servizi e alla magistratura. Ci hanno assicurato in questa circostanza una condizione ben diversa da quella vissuta da chi in quel tempo era anche presente nelle Aule parlamentari, quando, a metà degli anni '70, '70, di fronte alla prima insorgenza di manifestazioni terroristiche, tutte le forze politiche furono colte da smarrimento, cioè dalla difficoltà a capire e soprattutto a conoscere. Ma a capire e conoscere era anche impedito allo stesso Stato. Oggi vi è un punto positivo: le Forze di polizia e la magistratura, non dall'altro ieri ma dal 2004, hanno messo sotto osservazione, con i mezzi propri di una attività di polizia senza ricorrere ad altri strumenti impropri, le manifestazioni, le persone, le attività delle persone che hanno portato adesso a questo compendio conclusivo. La relazione del ministro Minniti sottintende una valutazione politica sulla quale occorrerà soffermarsi, e non soltanto oggi in questo dibattito, facendo proprie e riproponendo - lo aveva già fatto ieri Amato alla Camera - la

in primo luogo, abbiamo una riproposizione del terrorismo, quando credevamo, alla fine degli anni '80, che il terrorismo fosse debellato; ed anzi, debellato e superato con una ricomprensione politica da una parte - perché non riconoscerlo - con una politica del perdono che ha puntato al recupero. Anzi, ancora qualche mese fa abbiamo ascoltato - e sono tra coloro che non soltanto ascoltano questo discorso ma in qualche modo ne professano la convinzione - sull'esigenza di un superamento della stagione drammatica della democrazia italiana caratterizzata dal terrorismo. Ci troviamo in presenza tuttavia della permanenza e della riproposizione di questo fenomeno e abbiamo il dovere di fare delle analisi non di maniera. Senza dubbio, non occorre innanzitutto il minimalismo, che pure abbiamo constatato ieri e oggi anche su alcuni quotidiani di partito e alcuni quotidiani politici. Non occorre il senso discriminatorio della posizione tenuta da ambienti politici e giornalistici quando si deve prendere atto che l'obiettivo di questo gruppo terroristico era ben prefissato; e l'indicazione dell'obiettivo è già significativa del disegno politico che tale gruppo terroristico intende portare avanti. La solidarietà a Berlusconi, a Feltri, al professor Ichino, a «il Giornale» a tutte le possibili vittime designate, non può allora essere di maniera, deve anche implicare la consapevolezza politica che c'è qualcosa nel sistema politico, nel gioco e nel confronto politico che probabilmente va messo a fuoco in modo corretto.

Vorrei dire che lo stesso teorema Calogero, che non dovremmo dimenticare, anche perché potrebbe essere riproposto, coglieva questo aspetto essenziale proprio nella direzione della repressione di tutto ciò che a sinistra dell'allora Partito Comunista ci potesse essere, soprattutto in termini di dissenso radicale, di estremismo e, quindi, di violenza terroristica. Noi oggi, dopo 15 anni, abbiamo un sistema politico fondato sull'alternanza. Anzi, abbiamo provato e vissuto l'alternanza delle forze politiche. È vero, il sistema politico ancora non ha trovato il suo corso. Mi permetto un'osservazione che qualcuno potrebbe considerare fuori luogo: in una democrazia come quella italiana il sistema proporzionale è coessenziale alla democrazia, se vogliamo dare a qualunque dissenso una prospettiva diversa dal terrorismo. Ma qui ci troviamo di fronte ad un terrorismo che è ideologico, perché non riconoscerlo? Ed è un terrorismo ancora più pericoloso, perché si è proposto non la strategia combattente e militare ma la strategia dell'infiltrazione e della penetrazione. Ora, io rifiuto rifiuto i canoni ermeneutici dei comportamenti individuali o sociali in termini di responsabilità oggettiva, di responsabilità ambientale del «non poteva non sapere», che vanno però sempre Certo è che qui dobbiamo constatare che il livello, in cui questo fenomeno terroristico pensava e si proponeva di penetrare, era quello della CGIL. allora un problema del sindacato in Italia. Non per nulla abbiamo oggi una confluenza su un partito di centro-sinistra di tutti e tre i sindacati, e tuttavia è la CGIL, vittima, non sto dicendo altro, altro, della predestinazione di chi porta avanti un disegno terroristico. C'è allora una riflessione che anche i sindacati devono fare. Ho letto sui giornali di oggi le dichiarazioni del presidente Marini, che non può evidentemente ignorare o obliterare la sua grande responsabilità nella vita sindacale italiana, e questo è un richiamo che non può però risolversi in termini puramente predicatori, perché, al fondo di tale richiamo, c'è il limite che si deve dare al sindacato. Il sindacato in Italia, che per una certa stagione della nostra storia è stato anche positivo, non è stato soltanto soggetto sindacale, soggetto della contrattazione, è stato anche soggetto politico, perciò è stato predesignato nelle speranze dei rivoluzionari, di coloro che sognano la rivoluzione, ad essere lo strumento

sviluppate. Questa domanda politica, allora, non può rimanere inevasa. Il confronto politico e parlamentare, per parte nostra, sarà sempre estremamente responsabile, netto e alieno da ogni forma di strumentalizzazione. Ma su questo tema chi si ritiene erede del partito di Moro ha il dovere di essere rigoroso.

pronunciate parole nette di chiarimento che hanno contributo a ricondurre a maggiore tranquillità, diciamo nei termini giusti, il confronto politico su tale questione e, soprattutto,

per brevità e per non ripetermi faccio mie le parole in cui mi sono riconosciuta di più tra quelle già espresse, cioè quelle della senatrice Rubinato - nei confronti dell'operazione condotta e della procura di Milano. Credo non ci sia niente da sottovalutare e che tanto meno possa sottovalutare chi come me fa parte di una forza politica fortemente interessata a che tutte le espressioni del movimento, della protesta, delle lotte e dei conflitti si svolgano, abbiano possibilità di esprimersi e trovino sbocchi politici democratici. Anch'io voglio esprimere solidarietà piena, politica e anche personale a tutti coloro che sono stati individuati in questa operazione come obiettivi di di azioni criminali: il professor Ichino, il presidente Berlusconi, il direttore e la redazione di Libero, i direttori dell'azienda Breda, il dirigente della DIGOS,

Sono davvero felice, contenta - lo dico davvero senza alcuna retorica - di poter esprimere questa solidarietà in modo diretto perché, appunto, la prevenzione in questo caso è stata efficace.

Credo che bisogna capire di più come questi momenti, che poi sfociano nella piazza e nel ritrovarsi insieme in un luogo pubblico, provengono da percorsi, pratiche e idee della politica che sono radicalmente alternativi a quelli terroristici che vedono, invece, in queste forme forme qualcosa da colpire perché inefficaci, inutili a veicolare la protesta, il conflitto o, addirittura, perché sono forme di assimilazione nel sistema. Io credo - voglio essere molto chiara su questo aspetto parlando per il mio Gruppo politico - che sarebbe sbagliato se noi pensassimo (c'è qualcuno che lo pensa, troppi lo pensano) che una forza politica, un partito, una soggettività politica osta nelle istituzioni e nel Governo, osta nelle piazze, osta in quelle forme di pratica, osta in altre, nella politica che noi qui esprimiamo, nelle istituzioni. Credo che dividere, in primo luogo proprio noi, nelle persone che siamo, quello che qui facciamo (la nostra funzione di rappresentanza e di elezione politica) da quello che condividiamo con tanti altri uomini e donne che prendono parte a quella che si chiama la pratica dei movimenti - le pratiche sociali, direi in senso più lato - è qualcosa che contribuisce ad alimentare

prima di tutto perché vogliamo, perché lo facciamo parte di quel percorso e perché non riteniamo minimamente che ci aiuti a svolgere la nostra funzione - qui, nelle sedi istituzionali - perdere quel rapporto. Capiremmo meno, sapremmo meno, saremmo più separati. La rappresentanza non è mandato, non è solo delega; è relazione politica, è condivisione. Questa, come, Questa, come, in generale, le manifestazioni che nascono da ragioni vere e profonde di motivazione, di protesta ed anche di conflitto rispetto a scelte politiche fatte fatte dal Governo o comunque dalle sedi istituzionali non è mai solo contro. L'essere contro non vuol dire opporsi, negare, contrapporsi in modo frontale e verticale. Ogni manifestazione è anche un'espressione: per un diverso modo di intendere la questione, per una diversa maniera di individuare

Come forma - si chiedeva oggi Bocca, c'è un rischio costante di estremismo politico che sfocia nella violenza. Io credo ci siano delle ragioni da individuare oggi, nella fase politica e sociale in cui siamo, che non vuol dire cancellare una continuità ed un filo che ci lega agli anni '70. anni '70. C'è una società troppo frantumata, non sanamente divisa anche tra interessi, concezioni, idee (perché anche il conflitto di idee è un conflitto essenziale per la democrazia), - frantumata, fratturata. In questa frantumazione e in queste fratture ha preso piede, si è diffusa e troppo ha trovato spazio una cultura dell'odio sociale, del razzismo, del disprezzo, del rifiuto della differenza. Ne abbiamo sentito alcune espressioni anche in quest'Aula. Credo che un'altra ragione stia proprio nella semplificazione per non dire nell'impedimento della democrazia che - badate - è speculare a quello che il terrorismo propone. Come il terrorismo fa di un tutto Come il terrorismo fa di un tutto compiuto e omogeneo ciò contro cui combatte (lo Stato, il sistema, il capitale, usando le maiuscole) ed individua il bersaglio in un simbolo, in un uomo che

delega, a decisione, a potere e a chi ha il potere e anche alla personalizzazione. Una società destrutturata ed esposta alla precarietà chiede una politica che sappia essere invece l'elemento di strutturazione, di articolazione della società, di costruzione di rapporti, di sede di partecipazione, di protagonismo collettivo e condivisione.

solidarietà alle potenziali vittime, dal professor Ichino al presidente Berlusconi e al giornale «Libero». Consentitemi di aggiungere l'espressione della nostra solidarietà al vice questore questore della DIGOS di Padova, Pilleri, per quello che ha subìto questa notte. Il rigurgito del terrorismo interno non va sottovalutato. Serve una riflessione approfondita e senza strumentali polemiche, una riflessione culturale che coinvolga la politica, il sindacato e la società civile nella direzione dell'unità (abbiamo apprezzato questo passaggio dell'onorevole Minniti e cercheremo di dare il nostro contributo), unità che deve presupporre condizioni imprescindibili: la condanna del terrorismo e di ogni forma di violenza, nessun alibi che possa neppure larvatamente giustificare l'uso della violenza o la deriva terroristica. Nessun alibi, ripeto; e per evitare riflessioni sociologiche che ci porterebbero lontano e che appaiono a me stesso a volte fuorvianti, faccio un esempio concreto. C'è una legge sul lavoro e sul mercato del lavoro che qualcuno, nei luoghi di lavoro in genere, contesta perché, a suo modo di vedere, lo discrimina, lo precarizza. Costui ha pieno diritto alla protesta, ma quella legge e quel provvedimento non possono mai diventare alibi per giustificare la violenza o, peggio, l'organizzazione del terrorismo e gli atti conseguenti.

che la netta presa di posizione del segretario della CGIL, Epifani, in più interviste e dichiarazioni, è rassicurante perché è coraggiosa e va al cuore del problema. La CGIL si interrogherà e reagirà. Lo stesso Prodi oggi ha usato due termini dall'India: consensi e contiguità con il sindacato. Bene, la dichiarazione di Epifani e le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dall'India ci fanno fare un'ulteriore riflessione. Non ho però trovato accoglienza piena, e di questo mi rammarico ed esprimo tutta la mia personale preoccupazione e quella dei senatori di AN. Mi ha colpito, a tale riguardo (lo hanno ricordato altri, come poc'anzi ha fatto il collega Mannino), l'intervista del segretario della FIOM, Cremaschi, che pone gli accenti sul garantismo verso gli arrestati, al pari - dice - di quello assicurato a Berlusconi, più che sulla condanna netta al fenomeno che ci presenta. E quell'analisi accenna con toni giustificazionisti alle cause del nuovo terrorismo. Cito tra virgolette: «Esse trarrebbero giovamento» afferma Cremaschi «dalla solitudine di operai precari, dalle ingiustizie e dal malessere sociale. Non ci sono solo i precari ma tanti lavoratori a 1.000, 1.200 euro al mese che fanno una vita senza speranza, senza prospettive». Cremaschi dice poi di essere avversario dei terroristi, ma la sua analisi si tramuta ancora una volta nella ricerca dell'alibi, e questo non solo non è più condivisibile ma ci preoccupa molto, e auspico che preoccupi tutta quest'Aula. Così come occorre fare una riflessione sulla violenza negli stadi e fuori di essi. Quando un parlamentare dichiara che la morte di un giovane è uguale a quella di un poliziotto, *nulla quaestio*, dice una sacrosanta verità, ma dobbiamo andare al fondo del problema. Il poliziotto svolge il suo lavoro per consentire al giovane di poter manifestare in libertà o di poter assistere serenamente ad un evento sportivo. Diverso è l'atteggiamento di quel giovane che va alla manifestazione per spaccare le vetrine, per bruciare le auto e con le *molotov* in tasca. Con quest'ultimo non possiamo assolutamente essere clementi. C'è una differenza. Ma, tornando alle nuove BR, emergono aspetti inquietanti. Nell'ultima fase, prima di ritenere che lo Stato avesse sconfitto il terrorismo (c'è un passaggio della sua relazione, onorevole Minniti, che ci crea qualche difficoltà ad approvarlo, perché riteniamo che lo Stato purtroppo non aveva vinto contro le Brigate rosse), le Brigate rosse operavano in clandestinità. Nella nuova fase, vissuta solo pochi anni fa, a parte la brigatista Lioce, gli altri terroristi vivevano una vita normale: andavano a lavoro, rientravano in famiglia, frequentavano circoli sportivi. Oggi il fenomeno appare ancora più diverso: c'è un *mix* di vecchi arnesi del terrorismo e ciò dimostra che non era vero che erano state sconfitte le BR - e nuove leve, anch'esse apparentemente persone normali, e in più la presenza di giovani, troppi giovani. Occorre riflettere su quest'ultimo aspetto. Questi giovani come approdano al terrorismo? Da chi sono educati? Quali discriminazioni pensano di aver subito a vent'anni? In quale contesto hanno maturato tali convinzioni? Il più giovane arrestato è nato otto anni dopo l'assassinio di Aldo Moro. Insomma, cosa hanno visto? Possiamo liquidare il tutto con un semplice «perché sono dei delinquenti»? Credo che non lo possiamo fare. Dobbiamo tutti insieme analizzare ulteriormente questo aspetto. Poi torna la vecchia insoluta questione del sindacato, permeabile al fenomeno terroristico. Stime di questi giorni ci dicono che almeno 150 terroristi sono arrivati dal sindacato: perché? A me - ma non solo a me - pare evidente che costoro, più di essere contro il sindacato, intendevano occuparlo o comunque usarlo per destabilizzare le istituzioni, e forse nella loro follia pensano di poterlo ancora fare. Anche per questo abbiamo apprezzato le parole del segretario generale della CGIL, Epifani, così come abbiamo apprezzato che il segretario generale della UGL, Polverini, sindacato definito di destra e fino a poco tempo fa totalmente discriminato, soprattutto dalla CGIL, abbia espresso immediatamente solidarietà ad Epifani, compiendo un atto di grande civiltà. Per battere quindi il terrorismo occorre chiarezza e non mi pare che in queste ultime settimane la chiarezza politica sia stata presente nell'azione di Governo. Alcuni osservatori hanno messo in evidenza che la manifestazione di Vicenza non sia più del tutto estranea ai fatti di cui discutiamo. A Vicenza pare che non parteciperanno esponenti di Governo, bensì solo i dirigenti di tre partiti che fanno parte del Governo, due dei quali sono segretari nazionali; praticamente tre partiti decisivi, per la vita del Governo, manifestano contro il Governo stesso, praticamente quella parte che è a sinistra che dichiara di privilegiare l'ideologia delle poltrone. Massimo Franco ieri sul «Corriere della Sera» ha scritto. «Ma il doppio binario lascia margini inevitabilmente ambigui. Rifondazione che manda in piazza il gruppo dirigente, ma non le cariche istituzionali, è un concentrato di contraddizioni». Gli oltranzisti sostengono che è «una sceneggiata» e i più moderati richiamano al senso di responsabilità. L'ambiguità in politica è quasi sempre foriera di sbocchi totalitari.

dal SISDE due personaggi che da analisti avevano preparato l'operazione: appena avvenuta, sono stati cacciati; ci dovrebbe spiegare perché questo è avvenuto. In conclusione, vorrei ribadire che resto dell'idea che la politica, il sindacato e la società civile debbano fare muro, argine compatto contro la recrudescenza del fenomeno del terrorismo interno. Auspichiamo che nella sinistra si riesca a zittire e a e a isolare i giustificazionisti. E - me lo consenta onorevole Minniti - quando un segretario di partito dichiara che Berlusconi fa schifo questa è violenza verbale. Noi ci stiamo a lavorare con voi contro le Brigate rosse, ci stiamo ad un'operazione *bipartisan*, però, vi preghiamo, mettete ordine a casa vostra perché, quando un segretario di partito fa una dichiarazione del genere, certamente è difficile poter collaborare. L'unità di cui parlavo all'inizio dev'essere reale e fondata su princìpi e su presupposti comuni, senza sbavature e senza la ricerca ad ogni costo della causa che giustifichi la deriva violenta e la follia terroristica. La risposta che Alleanza Nazionale auspica dev'essere corale e deve coinvolgere le forze politiche tutte, il movimento sindacale tutto e la società civile. Fuori da questa possibilità ci sarebbe soltanto la confusione, la possibilità di creare *humus* su cui la violenza e il terrorismo possano annidarsi e riproporsi. Non voglio qui riprendere ciò che anche dei terroristi hanno dichiarato in questi giorni. Voglio soltanto concludere in questo modo: ringraziando il Governo ancora una volta per essere stato qui presente; e poi questa unità che oggi voi ci chiedete, perlomeno per quanto concerne gli aspetti del terrorismo, si può realizzare se al vostro interno l'ambiguità che ha serpeggiato in questi giorni, anche per la storia di Vicenza, viene meno. Senza ambiguità questa soluzione unitaria si può trovare.

A dispetto di quanti avevano preferito considerare la colonna brigatista Lioce-Galesi come una sorta di ultimo, disperato ed isolato gruppo crepuscolare, il fenomeno terrorista si è ripresentato con caratteri che lasciano intravedere una presenza diffusa di pulviscoli pronti a condensarsi in gruppi d'azione, cui si aggiunge una discreta dimensione di militanti antagonisti che giustificano e simpatizzano. Siamo ben lontani dalle forme organizzative degli anni di piombo, ma siamo altrettanto lontani dalla tesi di una patologia esaurita. Dopo la morte di Biagi, sollecitai vigilanza nel sindacato e nei luoghi di lavoro; ricevetti quale risposta un deciso rifiuto, perché fabbriche, uffici e sindacati erano puliti per definizione, anatemi e perfino una querela. L'Italia è l'unico Paese industrializzato ad avere avuto un persistente fenomeno terroristico ideologizzato per quasi quarant'anni. Come un fiume carsico, il terrorismo italiano, muovendosi con velocità, ampiezza e visibilità diverse nel tempo, proprio in ragione della sua radice ideologica, ha avuto costantemente due obiettivi privilegiati: il lavoro e l'imperialismo. Antony Giddens, il padre spirituale del *new labour*, ha recentemente detto dell'Italia: «Non conosco un altro Paese nel quale chi progetta una riforma del lavoro viene assassinato». Non solo Biagi, ma anche D'Antona, Tarantelli, Giugni, Taliercio ed altri ancora sono stati colpiti nel nome della distorta lettura del lavoro come fisiologico epicentro di un virtuoso conflitto sociale tra classi. Si tratta di una tesi sostenuta un modo delirante nei volantini brigatisti, ma che in forme appena più edulcorate si ritrova nei documenti di non piccole componenti sindacali e politiche nel nome di un mai ripudiato marxismo. Non si tratta di toni o di estetica del linguaggio, ma di analisi esasperate come quelle ancora presenti nel sito dell'ufficio giuridico della CGIL lombarda ove, a proposito della legge Biagi, si dice: «Un disegno autoritario nel metodo, eversivo nei contenuti». E se è accettato questo assunto, allora diventa comprensibile in alcuni la reazione violenta a questo disegno. La stessa considerazione vale poi per le persone oggetto di ricorrenti criminalizzazioni a sinistra, come fu per Marco Biagi, come è ancora - ieri - per Silvio Berlusconi. Non di meno l'imperialismo è stato la motivazione di altre azioni terroristiche, come il sequestro Dozier. Il clima creatosi intorno all'ampliamento della base NATO di Vicenza appare per questo pericolosamente idoneo a chi pensa di condizionare con l'azione criminosa la normale dialettica democratica. Onorevole Vice ministro, onorevoli colleghi, l'anomalia italiana è stata inevitabilmente - a nostro avviso - connessa alla presenza nel nostro Paese del più grande partito comunista dell'Occidente. Ciononostante, l'Italia non ha mai conosciuto quell'enfatica abiura del marxismo-leninismo che la socialdemocrazia tedesca ha deciso di compiere a Bad Godesberg. Ancora oggi, quindi, è essenziale che tutta la sinistra politica e sociale si ponga l'obiettivo del rifiuto esplicito di ogni base culturale della violenza politica e, in relazione a ciò, della riproposizione di un rigoroso confine a sinistra verso tutte le espressioni del radicalismo antagonista. Nella fase conclusiva degli anni di piombo - e purtroppo io li ricordo - fu certamente utile la linea del PCI allorché decise di segnalare tutto ciò che sapeva e di isolare con determinazione ogni forma di estremismo. Negli anni Novanta, tuttavia, la frettolosa e interessata rimozione del pericolo terrorista e l'affermarsi del confronto elettorale bipolare hanno fatto superare quel confine, nel desiderio di aggregare con colpevole superficialità tutto e tutti a sinistra. Non ci si stupisca poi se le indagini conducono ad inquietanti presenze nelle stesse organizzazioni sindacali. Questa inchiesta sarà davvero utile se concorrerà a rimuovere quel clima di giustificazionismo e perdonismo che ha portato perfino membri dell'attuale Governo ad ipotizzare atti di clemenza generalizzati e ha condotto molti ex brigatisti ed essere accettati financo come maestri di vita o consulenti di buoni sentimenti. Noi vogliamo concorrere a produrre una unità democratica contro il terrorismo affinché questa sia la stagione della sua definitiva rimozione, ma non possono non essere poste alcune condizioni per il superamento di questo clima: l'assunzione condivisa della «tolleranza zero» verso ogni forma di illegalità politica, dal vandalismo ai picchetti, al blocco di strade o ferrovie, l'erezione di un muro nei confronti di ogni forma di estremismo politico e sociale. Vicenza costituisce la prima occasione offerta alla sinistra politica e sociale per dimostrare la propria volontà e capacità di riproporre un rigoroso confine nei confronti di tutta l'area dell'antagonismo, che include quello strano simbolo del pacifismo violento e unilaterale, fenomeno ricorrente nell'esperienza italiana. La libertà di manifestare si coniuga necessariamente con la responsabilità delle grandi organizzazioni politiche e sindacali di governare la piazza, come hanno sempre saputo fare quando hanno voluto l'isolamento politico delle componenti più estreme. Il tema di Vicenza è quindi proprio questo: si vuole? Si vuole riproporre la fermezza della seconda metà degli anni Settanta, ora come allora non solo ovviamente verso il terrorismo, ma verso l'intera area a rischio, verso ogni forma di malattia infantile del comunismo, anche se ciò produce la perdita di segmenti di consenso nel nostro anomalo confronto bipolare? Come in presenza di un cancro del quale è impossibile conoscere la propagazione, l'intervento chirurgico deve essere significativamente più ampio rispetto al punto nel quale la malattia è accertata, in modo da isolare tutta l'area della possibile infezione.

che ha aggiunto qualcosa in più sulla manifestazione di sabato prossimo a Vicenza. Desidero spendere qualche parola sul punto. Vi sono due doveri in campo, in quella città, nella giornata di sabato. dovere è del Governo, ed è quello di garantire la libertà di manifestazione del pensiero di tutti coloro che andranno a Vicenza per protestare legittimamente in forme pacifiche; al tempo stesso, il Governo e le forze di polizia dovranno garantire la sicurezza della città.

in partiti della sinistra: essi devono isolare, condannare, bandire, escludere ogni forma di violenza, anche nelle parole d'ordine, anche nei simboli, perché è così che si rafforza la legittima protesta della città di Vicenza. Altrimenti, si fa il gioco di chi vuole soffiare sul fuoco.

che un'azione terroristica viene bloccata, neutralizzata, sconfitta, impedita prima che si realizzi con il sangue. quindi dobbiamo sottolineare che quei bersagli, i più ravvicinati, come anche quelli eventuali, possibili, sono stati protetti dall'azione congiunta del SISDE, della Polizia di Stato della magistratura di Milano. È stata così garantita la sicurezza di tutte le persone che erano, in diversa misura, a rischio ed in questo caso consentitemi di sottolineare che il capo dell'opposizione, l'onorevole Berlusconi, è stato efficacemente garantito nella sua personale sicurezza e nella sicurezza di una delle sue abitazioni, dall'impegno corretto e serio di magistrati quali il dottor Armando Spataro e la dottoressa Ilda Boccassini. paradosso agli amici che conoscono un po' di più le cronache giudiziarie, ma l'onorevole Silvio Berlusconi è stato protetto dal lavoro della dottoressa Ilda Boccassini. questi terroristi venivano da lontano, altri no: erano nuovi. E la serietà dell'inchiesta è intanto rivelata dal fatto che tre di loro si sono dichiarati prigionieri politici. Non credo sia in questo caso, sottolineare l'esigenza del rispetto delle garanzie e delle regole: sarebbe come sollevare un sospetto nei confronti dell'operato di quell'autorità giudiziaria, che invece lavora con correttezza e serietà. No, bisogna andare fino in fondo: la questione non è sollevare il richiamo del tutto ovvio alla presunzione di non colpevolezza; bisogna andare fino in fondo nell'accertamento delle responsabilità, nella individuazione dei complici, nella neutralizzazione di questo raggruppamento terroristico. Il dato su cui molti hanno proposto una riflessione, che dobbiamo compiere, è come sia avvenuto il reclutamento, perché vi siano giovani e giovanissimi accanto a vecchi dirigenti dei gruppi terroristici, che cosa giochi in questi giovani, cosa li spinga ad assumere simboli odiosi, che evocano soltanto sangue, miseria del Paese, lutti, divisione. È la rabbia? È la frustrazione? Dobbiamo riflettere su questo seriamente e vedo nel dibattito che è stato avviato tra le forze politiche una seria intenzione di riflettere e di agire insieme. Non posso non respingere il teorema proposto qui, ancora una volta, dal collega Sacconi, secondo il quale vi sarebbe una connessione ideale e culturale - questo è il punto la Confederazione generale italiana del lavoro, la FIOM e i gruppi terroristici, la sinistra politica, coloro che hanno alle spalle l'esperienza del Partito comunista di Enrico Berlinguer e i raggruppamenti terroristici: questo è un teorema che noi respingiamo. *(Richiami del Presidente)*. Ancora un momento soltanto, signor Presidente. Sappiamo fare le debite distinzioni, però, e siamo interessati ad un dibattito e ad un confronto unitario. Abbiamo apprezzato le parole misurate dell'onorevole Fini e, oggi, del senatore Matteoli, così come i giudizi preoccupati, ma seri e senza scivolate propagandistiche, dell'onorevole Casini e oggi, qui, del senatore Mannino. Le condizioni di un impegno unitario contro il terrorismo ci sono. Per quanto ci riguarda, consideriamo che si confrontano, che combattono battaglie nel rispetto delle regole, pacificamente,

nemici della sinistra, nemici dei riformisti. Noi dell'Ulivo richiamiamo come punti alti della ricerca dell'unità democratica in questo Paese i momenti nei quali la sinistra e i cattolici democratici erano insieme, nella linea della fermezza, come durante i giorni del sequestro Moro. I brigatisti sono nemici della democrazia e di tutte le forze che oggi intendano dare vigore e forza alla democrazia italiana, sia pure da posizioni contrapposte. Sono nostri nemici, li combatteremo fino all'ultimo respiro. un breve richiamo al Regolamento a conclusione di questa importante seduta. Mi riferisco, signor Presidente, agli articoli 23, comma 3, 40, comma 1, e 39 del nostro Regolamento. Ieri sera tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori della Commissione finanze e tesoro sul decreto-legge relativo alla direttiva comunitaria per Basilea 2, di fronte a un atteggiamento irresponsabile della maggioranza, che ha impedito perfino di correggere, lo sottolineo, macroscopici errori giuridico-formali. Crediamo che il Senato non possa essere considerato solo il luogo della ratifica di provvedimenti approvati dalla Camera. è, allora, un problema politico e regolamentare. All'articolo 40, comma 1, il nostro Regolamento prevede l'espressione di un parere obbligatorio sui disegni di legge

Ora, appare abnorme che su questo decreto non sia stato espresso il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea. Occorre una presa di coscienza del fatto che siamo fuori rotta,

ai vincoli di Maastricht e alle direttive comunitarie per non incorrere nelle infrazioni. Signor Presidente, le rivolgo un invito a far sì che almeno quest'Assemblea, quando martedì esaminerà il decreto-legge, possa avere contezza del parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Faccio appello, dunque, alla sua sensibilità affinché si faccia garante delle regole e quelle regole siano rispettate su questo decreto e sull'intero procedimento legislativo.

dibattuto di una posizione chiaramente strumentale da parte dei rappresentanti dell'opposizione, perché il percorso di approfondimento e di discussione previsto sull'oggetto era stato sviluppato in modo concertato in Commissione, con la messa a disposizione di un ampio spazio per la discussione, e nella sede di votazione sugli emendamenti e di valutazione dell'espressione del parere il relatore è stato puntuale nell'argomentazione di merito. Dopodiché, si può anche non essere d'accordo sul merito e sulle posizioni, ma questo non abilita nessuno ad affermare che vi è stato un atteggiamento irrispettoso da parte della maggioranza (mi pare davvero questa una forzatura interpretativa). Con riferimento all'elemento procedimentale, procedurale che

ma, ovviamente, ne ha molta meno nelle Commissioni, che sono le sedi di approfondimento e di discussione (che, molto spesso, vengono svolti anche con simpatia e con certo garbo).

emendamenti presentati dalle opposizioni, con fare sbrigativo sviluppa in pochissimi secondi il proprio parere, volendo appalesare una saccenza fuori luogo, non fa altro che produrre arroganza e mancanza di rispetto nei confronti di chi quel rispetto ha tenuto in conto svolgendo il proprio ruolo di opposizione e presentando, quindi, gli emendamenti che avrebbero potuto migliorare il testo. L'opposizione ha abbandonato i lavori, signor Presidente, in segno di protesta verso un comportamento inaccettabile che riteniamo abbia anche creato un imbarazzo al presidente al presidente Benvenuto, sempre accorto nei confronti dei diritti dell'opposizione. Non chiedevamo neanche rispetto da parte del relatore, perché questo significa ascoltare con l'intenzione di recepire quello che dice colui il quale parla; ma, almeno ci si aspettava un comportamento che facesse riferimento all'ottocentesca tolleranza nei confronti di chi, comunque, esercita

alle posizioni politiche. Abbiamo lavorato in Commissione: voglio dare atto sia al Presidente della stessa sia al relatore del provvedimento della correttezza e puntualità

merito del collega D'Amico sono state date con estrema puntualità e con dovizia di motivazioni e particolari, anche con un ragionamento interno, cosa che è naturale che avvenga, alla maggioranza. Ritengo che sia stata fatta una legittima scelta politica da parte dell'opposizione, ma una scelta tutta politica e tutta da giocare nella nella rappresentazione politica che con il merito delle questioni ha poco a che fare. È stato del resto comunicato ieri sera che che la scelta di abbandonare i lavori avrebbe dato luogo a una comunicazione esterna, a una conferenza stampa, cioè a un'utilizzazione politica dell'evento.

Cioè, il relatore studia gli emendamenti, comprende il contenuto normativo della proposta e su quello si esprime. Io ieri così ho ritenuto di fare, proprio in omaggio alla tradizione ottocentesca dei Parlamenti, secondo la quale il giudizio il giudizio - lo ripeto - entra sempre nel merito delle questioni. Comprendo che possa essere irritante il fatto che il parere del relatore fosse contrario, nel merito, su tutti gli emendamenti ma se il senatore Ventucci

la discussione entra sempre nel merito delle proposte normative, sia stato considerato addirittura uno sgarbo. Ho presente però molti casi (e il senatore Ventucci ne avrà presenti almeno tanti quanti me) nei quali è stata invece ritenuta e a me pare più giustamente, uno sgarbo un'opinione del relatore che si limitava ad esprimere pareri nella formula «sì» e «no», senza dare la spiegazione, dimostrazione della comprensione del contenuto normativo della proposta e la motivazione del proprio parere legata ai contenuti normativi stessi. per giustificare, ma forse per spiegare l'atteggiamento del Presidente della Commissione. Sono stato io che, guardando ai lavori di oggi, anche dall'esterno dell'Aula,